L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 7 maggio 2021 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze* «Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa

recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici",

Signor Presidente, devo informare l'Assemblea che ancora non siamo in grado di venire in Aula per discutere il provvedimento. Per terminare l'esame abbiamo bisogno di altre ore. Chiederei pertanto tempo fino alle ore 16 di questo pomeriggio.

tutta la contrarietà del nostro Gruppo per il modo di procedere nei lavori in Commissione e di conseguenza anche in Aula. È la seconda volta in due settimane che si verifica un inaccettabile ritardo nei nostri lavori, nostri lavori, dovuto chiaramente alle divisioni interne a questa maggioranza che si è messa insieme su presupposti che stanno venendo meno uno dopo l'altro.

Quindi, Presidente, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia annuncio una posizione molto dura su questo modo di procedere e non escludo che si possa arrivare anche all'occupazione dei banchi del Governo, se Governo e maggioranza

Presidente, anche a nome di L'Alternativa C'è esprimo contrarietà alla richiesta di sospensione. Non è possibile che in un momento come questo la maggioranza ritardi i lavori del Parlamento,

Presidente, il nostro lavoro ha fatto progressi. Purtroppo, però, non siamo ancora in grado di approdare in Aula. Pertanto, chiedo un differimento dell'arrivo in Aula del provvedimento a domani mattina, con la certezza di poter concludere i lavori in Commissione questa sera.

intanto - come si sa - la pazienza ha un limite. Quello che forse non si sa è che il limite è stato superato ampiamente e la pazienza è finita. Anche se siamo una opposizione patriottica e responsabile, sappia l'Assemblea che la pazienza è finita. Se è finita qui, dovete immaginare quanto sia finita fuori. Voglio ricondurre tutto alla realtà. Siamo stati convocati, dopo una Conferenza dei Capigruppo che ha approvato un calendario dei lavori all'unanimità la settimana scorsa, e abbiamo deciso che questa mattina avremmo

le misure di contenimento che da oltre un anno gli italiani, con molta pronta pazienza - quella che, appunto, è finita - stanno rispettando e anche patendo.

lavorato. Penso a tutti quegli italiani che stamattina sono andati regolarmente al lavoro e si chiedono perché qui non lavoriamo. Io dico che non ci fate lavorare, il che è un'altra cosa.

la questione è meramente politica. Quello che a Fratelli d'Italia preme sottolineare con chiarezza è anzitutto che qui si viene per lavorare e non per perdere tempo

quelle misure odiose che da oltre un anno condizionano la vita degli italiani: mi riferisco, tra le altre, al

il 15 maggio e riguarda le Universiadi di Torino; l'altra è il 17 maggio e riguarda la cabina di regia. Spesso e volentieri il Parlamento si sente mortificato, perché sostiene che il Governo decide e noi parlamentari non riusciamo a esprimere il nostro indirizzo.

che non contiamo niente e che nelle decisioni non ci siamo; ma se poi, quando c'è la possibilità di decidere, scappiamo, allora chi è causa del suo mal pianga se stesso. questa sarà la nostra posizione in Conferenza dei Capigruppo e sono convinto che la maggioranza abbia il dovere di trovare, con responsabilità e in modo maturo e non infantile, la mediazione sul tema delle riaperture.

della mozione stessa, questa venga stabilita dell'Assemblea del Senato. In particolare, l'articolo 55, comma 7, dice che «l'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda (...) di otto senatori, in relazione a situazioni sopravvenute e urgenti». A questo proposito ho qui pronta una mozione sulla questione della Guardia costiera libica, che sei giorni fa ha sparato ai nostri pescatori. Chiedo quindi che il Senato si esprima adesso, a fine seduta, per calendarizzare una mozione, sottoscritta

che molti difensori dei diritti umani ci dicono fare in realtà da carcerieri. Quindi, finanziamo i carcerieri dei migranti e, allo stesso tempo, con quelle stesse

Signora Presidente, come lei sa noi non siamo rappresentati nella Conferenza dei Capigruppo, quindi ci tengo a evidenziare anche il punto di vista sull'ordine dei lavori della costituenda componente L'Alternativa C'è.

questo stop, dovuto evidentemente alla mancanza di accordo in seno alla maggioranza, non comprima i tempi di discussione su argomenti fondamentali, in particolare sul tema delle riaperture e della riespansione dei diritti e delle libertà civili degli italiani, e che quindi

Chiedo pertanto che venga calendarizzata una discussione per poter dare al Governo indirizzi chiari per riaffermare le libertà di tutti i cittadini.

il calendario dei lavori sarà deciso in Conferenza dei Capigruppo, dove noi non siamo presenti. Le chiedo quindi di rispettare questo articolo, nel momento in cui viene avanzata Fattori, intanto le chiederei il testo della mozione con i proponenti.

trovo abbastanza imbarazzante dover sospendere una discussione che incide su un tema attuale come quello dei

un timore, cioè quello di apparire soggetti di una sperimentazione. Io avrei voluto che nel corso della discussione del decreto-legge si facesse anche riferimento a questo, perché è importante.

attualità. Non capisco il motivo per cui si continui a rimandare la discussione. Evidentemente lo scollamento dentro la maggioranza è tale che il Paese va

Senatrice Fattori, abbiamo avuto qualche minuto per poter verificare e capire meglio i termini della sua richiesta. È corretto ciò che lei ci ha chiesto anche ai sensi dell'articolo 157

La contestualità non arriva al punto che lei possa direttamente portarlo in Aula senza l'acquisizione e la pubblicazione. Per

Spero di essermi spiegata. Lei ha ragione nell'appellarsi all'articolo che ha indicato, ma manca un presupposto. manca un presupposto. Ho capito che è un argomento cui lei giustamente tiene. Avrà sicuramente modo di presentarlo in maniera tale che possa essere perlomeno preso in considerazione. Se, come ritengo, sono terminati gli interventi sull'ordine dei lavori, come preannunciato, sospendo la seduta,

saranno discussi il decreto-legge sul contenimento dell'epidemia Covid-19, vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici, nonché le mozioni sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19 e sulla candidatura di Torino alle Universiadi del 2025. Al fine di concludere l'esame dei predetti provvedimenti nella giornata di domani, si è proceduto alla riduzione dei tempi assegnati il 6 maggio scorso per la discussione generale del decreto-legge. Si è altresì convenuto che la discussione delle mozioni sulla candidatura di Torino alle Universiadi del 2025 sia limitata alle sole dichiarazioni di voto, della durata di cinque minuti. Il *question time*, già previsto per le ore 15 di domani, non avrà luogo. La Conferenza dei Capigruppo è convocata domani, alle ore 12,30, durante la sospensione della seduta per la sanificazione dell'Aula, per stabilire il calendario dei lavori delle prossime settimane. Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la seduta di costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare

Signor Presidente, signori senatori, oggi, nella Giornata internazionale degli infermieri, sento il dovere di rivolgere loro tutta la mia gratitudine per l'impegno a cui sono stati chiamati in questi duri tempi di pandemia. La data del 12 maggio è stata scelta in occasione dell'anniversario della nascita di Florence Nightingale, considerata la madre dell'infermieristica moderna. A lei dobbiamo l'applicazione del metodo scientifico all'assistenza medica. Fu una donna iconica, che spese la sua vita nella cura dei malati con professionalità e dedizione, nonostante fosse affetta da fibromialgia, che le causava grandi sofferenze. Infatti oggi in suo onore ricorre anche la Giornata mondiale per la fibromialgia, una sindrome tutt'altro che rara, che coinvolge circa due milioni di italiani. Da tempo mi interesso al tema; ho depositato il disegno di legge n. 899, affinché la fibromialgia sia riconosciuta come malattia invalidante a tutti gli effetti. La fibromialgia è purtroppo una patologia ancora poco conosciuta e la scarsa diffusione di informazioni rende la diagnosi molto spesso estremamente difficile; questo fa sì che le persone affette da questa malattia non riescano a ricevere cure adeguate in tempi brevi, perché spesso si hanno difficoltà a riconoscere i sintomi e a comprendere che la patologia è la causa del dolore. dolore. Oltre alla malattia, queste persone scontano un senso di isolamento, che causa ulteriori sofferenze. Per questo motivo, credo fermamente che dare visibilità a questa patologia e ai suoi sintomi possa aiutare concretamente milioni di persone in Italia e nel mondo. Ringrazio l'associazione Libellula Libera, con cui ho avuto modo di collaborare in questi anni e a cui va tutta la mia stima per il lavoro quotidiano che svolge. Colgo l'occasione anche per ringraziare sentitamente il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, per aver reso possibile illuminare oggi di viola Palazzo Madama. L'iniziativa è stata promossa dalle associazioni più rappresentative di pazienti fibromialgici ed è stata accolta da molte amministrazioni, che questa sera illumineranno di viola piazze e monumenti in tutta Italia. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni dei pazienti affetti da fibromialgia, ma anche di diffondere maggiore conoscenza e promuovere la prevenzione. Indossare oggi un fiocco è un piccolo gesto che può significare tanto per tantissime persone. Io lo farò, insieme ai miei colleghi, nella speranza che siano in tanti a seguire il nostro esempio. Illuminiamo la fibromialgia per non lasciare nell'oscurità il dolore di tanti pazienti e delle loro famiglie.

la fibromialgia come una malattia e colgo l'occasione per dire che vi è un disegno di legge che giace da moltissimo tempo in Commissione sanità

hanno bisogno di avere questo riconoscimento. Non devono essere invisibili, dobbiamo renderli visibili, devono avere dei punti di riferimento, ci devono essere i centri di riferimento regionali: questi

come spesso capita in questi casi. Quando non ci sono le risposte da parte del Servizio sanitario nazionale, purtroppo accade che altri spaccino come efficaci cure che non lo sono, quindi si pone anche un problema di legalità.

Signor Presidente, vorrei far presente una situazione che mi è stata sollecitata dalla categoria del *wedding*, cioè delle cerimonie per matrimoni,

musicisti e tanti altri, che stanno chiaramente patendo la situazione di chiusura, tra l'altro con l'impossibilità di programmare, non avendo indicazione di una data di inizio

è anche per le giovani coppie che desiderano convolare a nozze, cui potrebbe permettere una programmazione più serena. Alcune coppie lamentano anche il fatto di avere più volte posticipato la data. Questo particolare non è relegabile al

e degli eventi, chiede l'indicazione di una data certa ed inequivocabile di desidero porre all'attenzione dell'Assemblea l'inverosimile vicenda di Lara Lugli. Lara è una pallavolista, la cui squadra, l'Associazione sportiva dilettantistica Blu Volley Pordenone, militante in serie B1, fece firmare due anni fa una scrittura privata con relativo accordo finanziario, in cui era presente, nero su bianco, una clausola anti maternità, ossia un articolo per cui la gravidanza era motivo di risoluzione dell'accordo stesso. Nel 2019, verso la fine della stagione sportiva, Lara si scoprì incinta e la Volley Pordenone la licenziò, senza nemmeno pagarle l'ultimo mese di attività. Un mese più tardi perse il bambino, a causa di un aborto spontaneo, ma la *querelle* con la dirigenza si ripresentò due anni dopo, quando Lara venne citata per danni, rea di aver compromesso la stagione della squadra con la sua gravidanza; ciò in risposta - che non esito a definire intimidatoria - a una sua ingiunzione ingiunzione relativamente al mancato pagamento dello stipendio di febbraio. Circa due mesi fa la giocatrice ha denunciato tutto pubblicamente e, oltre al clamore in Italia, la notizia dell'accaduto è stata rilanciata dal «New York Times» e dal «The Guardian». Secondo quanto dichiarato dalla stessa Lara, l'atleta avrebbe dovuto informare la dirigenza dell'eventuale desiderio di gravidanza. A sostenere la sua causa sono intervenute l'Assist, l'Associazione nazionale atlete, e l'Associazione italiana pallavolisti, chiedendo che la citazione venisse ritirata e che Federvolley e CONI prendessero provvedimenti nei confronti della società sportiva, cosa che ad oggi non è avvenuta. Sul caso è intervenuta anche la presidente Alberti Casellati, che ha dichiarato: «Invocare la condanna della pallavolista Lara Lugli perché in maternità è una violenza contro le donne. La maternità ha un insostituibile valore personale e sociale». A nome del MoVimento 5 Stelle chiediamo alla ministra Bonetti e alla sottosegretaria Vezzali (una sportiva, tra l'altro) di dimostrare pubblicamente la solidarietà dei vertici dello sport italiano a una donna che ha visto negato il proprio diritto di essere madre e a ricevere le conseguenti tutele. Il prossimo 18 maggio Lara dovrà andare in tribunale da imputata, solo perché incinta a trentotto anni. La ritengo una offesa a tutte le donne e alle atlete italiane, oltre che al nostro Paese e allo sport italiano. quindi, che il Governo mostri concreta vicinanza a Lara Lugli e, nel rispetto dell'autonomia sportiva, chieda chiarimenti ai vertici di quella Federazione e al Comitato olimpico nazionale.